L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 1905, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»,

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - sull'emendamento 12.0.300 parere non ostativo, segnalando la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti legislativi ivi previsti; sull'emendamento 14.0.300 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare il pieno rispetto delle competenze regionali nella definizione della disciplina organica della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale Specialista; - parere non ostativo sui restanti emendamenti». parere non ostativo sui restanti emendamenti». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

del 2010"; - che all'articolo 14, comma 3, lettera *e),* dopo le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica" siano aggiunte le altre: "ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei" e che siano soppresse le parole: "o rimborsi spese". Il parere non ostativo è reso nel presupposto che l'inclusione tra le erogazioni liberali a favore delle università, di cui all'articolo 4, comma 9, anche quelle a favore del "Fondo per il merito" non determini effetti di riduzione del gettito considerando l'effetto di sostituzione che si determinerebbe tra le erogazioni a favore delle università. Il parere non ostativo sull'articolo 9 è reso nel presupposto che, stante la variabilità delle risorse del Fondo per la premialità, le prestazioni da esso erogate siano temporanee in relazione alle risorse disponibili».

Presidente, rispondo al senatore Rusconi che il Ministero si sta impegnando per trovare altri fondi a sostegno della riforma, per cui la raccomandazione ha una grande valenza politica in questo senso.

portano nel testo quanto stabilito dalla Costituzione stessa, vale a dire che le competenze in materia di diritto allo studio sono esclusivamente delle Regioni. pertanto, non deve operare in "armonia" con le Regioni, ma "nel rispetto" delle competenze delle Regioni stesse. Il Governo può e deve stabilire i livelli essenziali delle prestazioni per quello che riguarda il diritto allo studio ed erogare i finanziamenti conseguenti per coprire integralmente quei livelli essenziali, secondo quanto stabilito dalla legge sul cosiddetto federalismo fiscale, la n. 42 del 2009. Si tratta

anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Nello stesso articolo 34 poi, all'ultimo comma - con una norma secondo me molto puntale, ma, proprio perché così puntuale, indicativa di una priorità individuata dalla Costituzione stessa - si stabilisce: «La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze». Dunque la Costituzione dà indicazioni molto precise sul diritto allo studio che riguardano borse di studio, servizi per gli studenti, trasporti, alloggi, collegi, biblioteche, sale studio,

che svilupperemo meglio nella discussione relativa all'articolo 4, intitolato al fondo per il merito. È indispensabile che le provvidenze per premiare i meritevoli siano collegate a livelli di reddito insufficienti per percorrere adeguatamente il percorso scolastico.

Il diritto allo studio costituisce proprio questo insieme di provvedimenti di accompagnamento. fare una gara può essere anche una cosa positiva, ma il tema è questo: non si può gareggiare e fare un medesimo percorso con una bicicletta o con una motocicletta; coloro che sono in possesso della motocicletta, anche se sono molto meno bravi e molto meno capaci di coloro che corrono in bicicletta, arriveranno sempre primi. È compito della Repubblica dare a tutti lo stesso strumento per gareggiare. Quindi, chiedo che questo principio

La seduta è ripresa.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 1 a 7, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.304, 1.307, 1.0.303,

3.0.300, 3.304, 4.304, 4.305, 4.314, 5.306 (limitatamente alla lettera 5.318, 5.0.300, 6.300 (testo 2) (limitatamente alle lettere *g)* ed *h*), 6.301, 6.0.300 7.301, nonché parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.317 (testo 2), 2.309 e 2.310. Esprime poi parere non ostativo reso, ai sensi della medesima norma costituzionale, alle seguenti condizioni: - che alle proposte 2.302 (limitatamente al capoverso 2.303 (limitatamente alla lettera *f*) e 2.353 siano aggiunte in fine le seguenti parole: "La partecipazione all'organo collegiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese"; che al comma 6 dell'emendamento 4.1 le parole: "non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro" siano sostituite dalle altre: "non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro". Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7».

1.301. L'emendamento 1.302 è sostituito dal testo 2, su cui si esprime parere favorevole.

1.308 ritengo che la formulazione adottata in Commissione sia ancora più forte e più garantista rispetto alle esigenze espresse espresse dalla senatrice Bastico in confronto all'introduzione del termine «ancorché»; infatti si esclude che coloro che non siano privi di mezzi possano usufruire di questo tipo di borse di studio.

Signor Presidente, il nostro Gruppo ha inteso sottolineare che le università sono sedi primarie di libera ricerca e libera formazione, ma sono anche sedi pubbliche di libera ricerca e libera formazione. L'emendamento 1.300, che noi sosteniamo, tende a sottolineare la dimensione europea dell'università, che deve essere inquadrata nell'ambito di tutte le politiche tendenti a rendere attrattivi i nostri atenei, rispetto soprattutto al conseguimento di politiche di implementazione di tutto il triangolo della conoscenza, obiettivi di sviluppo e innovazione, che in questa legge sembrano essere presenti.

in quanto garantisce l'utilizzazione di parametri di efficienza e di trasparenza che sono comuni a tutto il territorio nazionale e a tutto il sistema e riesce a favorire anche l'organizzazione privata in una dimensione più rafforzata rispetto alla missione istituzionale dell'università. Questo è il senso della nostra proposta e riteniamo che un Governo che porta avanti un disegno di legge come questo, ancorandolo al merito e ad una serie di innovazioni che sono anche importanti, non possa non avallare

Signor Presidente, invito i colleghi a sostenere il nostro emendamento, volto all'inserimento di una definizione di università più ampia in riferimento al concetto di elaborazione e circolazione della conoscenza da specificarsi meglio nella formulazione proposta; essa contiene infatti un riferimento diretto all'apprendimento ed alla elaborazione critica della conoscenza e non alla sua circolazione.

non si fa affatto riferimento alla necessità che la valutazione dei risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca delle università

Questo è un tema cruciale perché la natura di terzietà dell'Agenzia di valutazione è condizione importante per poter introdurre elementi di valutazione oggettiva della qualità. Anche nel lavoro della Commissione un miglioramento al testo del disegno di legge concerne proprio, in molti passaggi, la specificazione della funzione e dell'importanza dell'ANVUR proprio a garanzia della qualità della valutazione. Questo è un tema che, perlomeno, rispetto alle università eccellenti, ripristina quei principi di autonomia, di responsabilità, di valutabilità e di conseguenza di meritocrazia che a più riprese ho avuto modo di sostenere e che sono stati posti alla base della filosofia di questo disegno di legge, ma poi in smentiti in molte circostanze dal testo.

visto che l'ANVUR sarà composta da esperti nazionali e internazionali di altissimo livello. Ci sembra una proposta che rispetta quei criteri di merito, di valore e di eccellenza che il Ministro ha richiamato ieri. Un po' di coerenza ogni tanto vorremmo che ci fosse!

di fatto condiziona il diritto costituzionale all'autonomia, previsto dall'articolo 33 della Costituzione, alla virtuosità di bilancio:

Fra l'altro, viene meno quel principio di responsabilità per cui il Governo dovrebbe invece invitarle, nella loro responsabilità e nella loro autonomia, a diventare virtuose. È come se non si riconoscessero dei diritti fondamentali

vorrei invitare il senatore Procacci a rileggersi attentamente la Costituzione, che parla di autonomia nei limiti previsti dalla legge. La legge, quindi, prevede dei limiti stringenti proprio per garantire che questa riforma importante della *governance* sia fatta per raggiungere risultati di maggiore efficienza e non invece per consentire di svicolare rispetto a prescrizioni normative.

del testo è sostenere effettivamente quelle realtà che hanno dei problemi territoriali, ma hanno altresì anche un elevato valore culturale che, altrimenti, non potrebbe essere sostenuto. Però così non è scritto, così non è specificato. Parlando cioè di università svantaggiate non si capisce bene a che cosa fa riferimento la norma e come si possa applicare; peraltro, essa sembra di fatto implicare un aiuto da parte del Ministero. Il sistema, a nostro avviso, deve poter mantenere una sua coerenza tenendo conto dei meccanismi di valutazione, e l'unico modo per poter evitare che criteri standard di valutazione possano compromettere università che hanno un elevato valore culturale per il territorio è prevedere, in sede di criteri di valutazione, che si dovrà eventualmente tener conto di fattori relativi al contesto territoriale e socio-economico per evitare che venga compromessa la valutazione dei risultati conseguiti. Relatore Valditara, mi appello anche alla sua competenza in merito. Parlare di università svantaggiate senza specificare ulteriori qualificazioni di questo concetto ci sembra effettivamente molto pericoloso e può aprire la strada a considerazioni che non sono assolutamente condivisibili. Per

su base interregionale (ad esempio, tra il Piemonte orientale e l'Insubria evitando ad entrambe di cadere nelle fauci, rispettivamente, di Torino e Milano) e non solo su base regionale. Anzi, personalmente auspico che possano essere stipulati persino accordi di programma tra università transfrontaliere: penso all'università della Svizzera italiana per la Lombardia, alle università svizzere e francesi delle regioni confinanti con il Piemonte, all'università di Mentone per la Liguria, all'università dell'Austria per il Trentino-Alto Adige, e così via. L'emendamento per un verso limita la possibilità per alcune grandi università di fare la voce grossa, atenei che nella qualità di capofila si sentono legittimati a chiudere sedi secondarie aperte con tanti sacrifici dalle istituzioni locali, quali le Province, i Comuni, le fondazioni e le camere di commercio, per razionalizzare i costi. cito il Politecnico di Torino, che non ha avuto remore a chiudere la sede di Vercelli - pur contando 1.000 iscritti ed avendo tante risorse messe a disposizione dagli enti locali per portare a Torino gli studenti che, magari, avrebbero potuto guardare a Milano con un accordo di programma interregionale al fine di salvare l'ateneo, tanto caro alle istituzioni della provincia di Vercelli e dintorni. Per altro verso, si dà la possibilità alle università

"*performance*" e sostituirla con la parola italiana "risultati" sia giusto e naturale. Questo interpella, tuttavia, un problema che riguarda anche gli uffici - se posso permettermi - del Senato e del Parlamento, e cioè l'abuso

in lingua inglese, che accettiamo di inserire nel nostro ordinamento per pigrizia. Non credo che si debba chiedere un parere all'Accademia della Crusca

un parere per sfrondare, trovando non dei sinonimi ma le appropriate parole in lingua italiana con le quali gradualmente sopprimere le superflue parole in lingua inglese che abbiamo introdotto nel nostro ordinamento. *(Applausi

non solo la difesa di un'identità linguistica e culturale, ma anche un problema di comprensibilità delle norme e delle leggi. In questo caso, trattandosi di una legge relativa all'università, alla cultura e all'identità culturale del Paese, più ancora che per altre leggi mi sembra che l'osservazione del senatore sia giusta e fondata. Il nostro

Se ha senso italianizzare un documento fondamentale come questo, posto che si può essere anche contrari, è inutile cambiare l'unica parola che anche in italiano si capisce*.* "*Tenure track*", da una parte, e, sicuramente, "*governance*",dall'altra, sono termini molto più complessi, e quindi occorrerebbe non soltanto ripulirli

dal provincialismo in cui la nostra università è piombata ormai da troppo tempo, anche l'assunzione di un vocabolario un po' più ampio, senza fare alcuna offesa alla nostra lingua madre, che possa avere una capacità di essere compreso anche da studenti che non sono italiani, forse non è così scandalosa come possiamo oggi sostenere.

occorrerebbe sopprimere la dicitura "risultati" e inserire quella di "prestazioni" o analoga, altrimenti rischiamo di vincolare ai risultati

quindi, i colleghi ad andare al sodo: qui si parla di riformare l'università e non di riformare il vocabolario. Questa è un'altra cosa!

un finanziamento dovuto al sistema dell'alta formazione universitaria in questo Paese per fare decollare le nostre università, farle uscire dal provincialismo e renderle competitive,

era assolutamente ovvio e necessario, Ministro, che il coraggio si spingesse oltre l'ostacolo: vale a dire, bisognava abolire il valore legale del titolo di studio. Il valore legale del titolo di in una certa materia, come se i percorsi formativi fossero tutti uguali e fossero tutti arrivati ad una soglia accettabile - non elevatissima, né elevata - di valore culturale. Così sappiamo che non è.

su questa riteniamo che il coraggio da lei dimostrato altre volte debba spingersi oltre l'ostacolo. Abbia il coraggio di farlo: effettivamente renderemo un grande servizio al nostro sistema formativo universitario, a quello di eccellenza, e ai nostri giovani che potranno competere con le armi della competenza e della cultura

Il nostro sistema universitario ha 60 università statali, 17 non statali legalmente riconosciute, sei istituti superiori ad ordinamento speciale e 12 università telematiche. La legge n. 133 del 2008 ha previsto una sostanziale e drastica riduzione delle risorse e dei finanziamenti al sistema universitario, in particolar modo al Fondo di funzionamento ordinario, prevedendo un taglio di 63,5 milioni di euro per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni di euro per il 2011, di 417 milioni di euro per il 2012 e 455 milioni di euro per il 2013. Parliamo complessivamente di circa un miliardo e mezzo di euro di riduzione in cinque anni, pari ad una media di 300 milioni di euro in meno ad anno:

Se guardiamo poi al dato della spesa annuale per studente, risulta che l'Italia è all'ultimo posto dopo gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, la Francia la media OCSE è di 11.512 dollari a studente, noi siamo ad 8.026 dollari. Se guardiamo alle retribuzioni dei docenti italiani, sono tra le più basse

drastica il sistema dell'università. Quindi, il testo che abbiamo davanti più di quello che scrive non può scrivere: è ovviamente limitato anche dalla circostanza (lasciando stare che il sistema della valutazione dell'università sta fuori)

rivoluzionare il sistema della formazione e dell'offerta universitaria, affidandola al mercato (nel senso buono del termine) e alla scelta di qualità che gli studenti e le famiglie italiane fanno rispetto ai singoli atenei: tutto ciò nel momento in cui cade il monopolio statale del titolo di studio. Forse questo è il modo migliore per contrarre il numero delle università e soprattutto per andare a «cecchinare» quelle università che sono improduttive - che stanno al Nord e al Sud del Paese del Paese - e superfinanziate (pubbliche o private che siano) in modo da far selezionare agli studenti come e dove fare la formazione universitaria per il futuro. Questo è il senso della nostra proposta e per questo riteniamo che sia impossibile cavarcela con un ordine del giorno che potrebbe anche togliere dall'imbarazzo - ce ne rendiamo conto - una parte della maggioranza che sta discutendo al suo interno su questo tema. Ci sono stati interventi sulla rivoluzione liberale del sistema universitario che ruota attorno all'abolizione del valore legale del titolo di studio. Vediamo se questa anima liberale del centrodestra esiste e se ci dà una mano a sostenere anche questi emendamenti.

luogo perché, nei cinque mesi di discussione in Commissione (ne sono testimoni i

un emendamento in Aula, estrapolandolo da una discussione che è durata cinque mesi. In esso si parla della «previsione di accesso automatico alle professioni», mentre quest'Aula sta discutendo ad esempio dell'ordinamento della professione forense.

specie per chi ha interessi plurimi, non vedo perché non si possa arrivare in Aula con proposte che tra l'altro non sono formulate *ex abrupto*, dato che se ne è già parlato, almeno in questa legislatura, un paio di volte. Tenuto presente anche ciò che il relatore ha incluso nella propria replica

tenuto conto anche dei tempi necessari per una riforma che, come ricordava poco fa la senatrice Sbarbati, è radicale ed è l'unica che può finalmente mettere la nostra università alla pari di quelle europee e del resto del mondo, a cui guardiamo come modello. Pertanto, anche a nome della senatrice Poretti, dichiaro che voteremo a favore di questo emendamento

Presidente, fermo restando che ognuno si deve sforzare per quanto possibile di partecipare ai lavori sia delle Commissioni che dell'Aula, mi pare che sul piano del metodo sia di buon senso, oltre che di buon gusto, la considerazione di chi mi ha preceduto. Non vedrei questa strettissima connessione fra l'abolizione del valore legale in tutte le scuole

separata dalla responsabilità. Se vogliamo procedere verso una combinazione di autonomia e responsabilità,

è un invito a trasformarlo in ordine del giorno.

autonomia di gestione nell'ambito di specifici criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a)*»*.* Chiedo quindi al senatore Calabrò se è disponibile ad accettare questa riformulazione.

una soluzione potrebbe essere, per esempio, quella di immaginare una votazione congiunta di senato accademico e consiglio di amministrazione. Ritengo però che sia preferibile concordare una soluzione che credo possa coinvolgere maggioranza e opposizione.

al comma 1 dell'articolo 2 sia detto che «nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione» gli statuti dei singoli atenei disciplinino l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, tutto quanto può essere stabilito dall'autonomia dello statuto sia di competenza degli atenei. Parliamo tanto di autonomia: lasciamo fare agli atenei! In questo disegno di legge c'è già troppo, sono addirittura delineati contratti di lavoro, il che non è proprio di una grande riforma dell'università: lasciamo più respiro all'autonomia degli atenei. Penso che aggiungere questo in premessa e dare maggiore libertà ed autonomia

Ho già mandato la senatrice Mongiello a ritirare la scheda.

rendere più chiara la differenza, assai ambigua invece nel testo, tra senato accademico e consiglio di amministrazione. In ogni apparato di qualche complessità, come è noto, se non si rendono evidenti i compiti, si creano situazioni assolutamente anomale: conflitti di competenza o ingerenze improprie in compiti che non spetterebbero a quell'organismo. Per esempio, cito un caso per tutti: nel testo si attribuisce al consiglio di amministrazione, impropriamente, la competenza di deliberare sull'attivazione o soppressione di corsi e dunque dunque questo, che è un tipico aspetto inerente all'indirizzo didattico, pedagogico, culturale, viene sussunto dall'organismo di amministrazione in un non detto che corre come sottotesto in questo disegno di legge, cioè che si vorrebbe aziendalizzare l'università. In verità non si aziendalizza nulla perché è tutto tagliato; però rimane l'ideologia dell'aziendalizzazione. E questo è un punto

il presente emendamento che abbiamo presentato su proposta del CUN è volto a meglio specificare le modalità di elezione del rettore, allargando la platea dei soggetti che potranno partecipare alla votazione. Noi riteniamo utile per una maggiore democrazia coinvolgere al voto tutto il personale che opera nelle università, come i docenti ricercatori, il personale tecnico-amministrativo ed i rappresentanti degli studenti,

delle risorse che il consiglio di amministrazione fissa in materia di didattica e di ricerca. La competenza principale e più importante deve però restare, secondo noi, al senato accademico.

Signor Presidente, visto che il senato accademico è l'organo competente a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, con l'emendamento 2.319 si chiede che esso sia composto in materia prevalente dai direttori dei dipartimenti,

è di tutta evidenza che loro la pensano in modo opposto e contrario. La maggioranza e il Governo sostengono cioè che il consiglio di amministrazione di una università, oltre ai compiti tipici e ampi che noi descriviamo, di gestione, amministrazione e strategie in termini finanziari, abbia anche funzioni strategiche rispetto alle finalità accademiche. Francamente, l'università non ha compiti mercantili. Una buona gestione appartiene a tutte le istituzioni e a tutti gli organismi, è doverosa, ma le funzioni di un consiglio di amministrazione rispetto ad un senato accademico devono essere diverse e distanti, per evitare che anche all'università possano esserci delle cricche. in tale emendamento, purtroppo seguendo la logica prescrittiva di questa legge, qual è il numero massimo degli esterni che vi devono partecipare, perché prevedere, come era all'inizio,

chiarezza, trasparenza, valutazione del merito, finanziamento adegua, deve rientrare anche una distinzione di compiti fra ciò che è gestionale e ciò che è strategia accademica.

un'appropriatezza adeguata ai tempi, che oggi la richiedono sempre più lunga e sempre più approfondita. Faccio voti affinché il Governo

di amministrazione. Tra l'altro, in Senato sono stati depositati altri disegni di legge che prevedono questo, ad esempio per le società quotate in borsa e per altri organismi. Io stessa sono presentatrice di un disegno di legge che va in questo senso. Invito la signora ministro Gelmini,

una risposta concreta al problema della sottorappresentanza delle donne nei consigli d'amministrazione, cioè nei luoghi in cui si decide. Ripeto: le università avrebbero tutto da guadagnare da una rappresentanza delle donne superiore a quella attuale.

Presidente, l'emendamento 2.330 punta semplicemente a prendere sul serio il ruolo che il Governo vuole attribuire al consiglio di amministrazione. un normale consiglio di amministrazione fosse dichiarato lo stato di dissesto sarebbe bene che si sciogliesse. Mi sembra una cosa elementare: è un modo di prendere sul serio le intenzioni del Governo.

anche questo emendamento è volto all'inserimento di limiti all'operato del direttore generale, il quale nel dirigere i servizi dovrà tener presenti le indicazioni rivoltegli da tutti gli organi previsti al comma 1 del medesimo articolo, ovvero il rettore, il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Pertanto invito i colleghi a sostenere questo emendamento e

**Il Senato non approva**.

**Il Senato non approva**.

Prima abbiamo persino bocciato il fatto che l'ANVUR possa valutare l'eccellenza di alcune università e che queste, a loro volta, possano derogare rispetto al modello di gestione e organizzazione di ateneo.

di sviluppare il merito delle proprie competenze in materia di ricerca, oltre che in materia di organizzazione della didattica dei dipartimenti. Che bisogno c'è? Insomma, questo Governo ha istituito per la prima volta un Ministero del federalismo, e qui non si riconosce autonomia; ha per la prima volta un Ministero per la semplificazione, e qui si complica burocraticamente la vita degli atenei.

Ma questo contraddice il fronte della ricerca di moltissimi dipartimenti: pensiamo solo che molti premi Nobel vengono attribuiti a scoperte negli spazi cerniera e al fatto che un dipartimento di neuro-psico-immunologia non si potrebbe mai fare. cadere l'omogeneità delle afferenze scientifico-disciplinari, per favorire la creatività e il merito della ricerca. È la dimensione transdisciplinare e interdisciplinare che caratterizza la frontiera della ricerca in quasi tutti i campi: per quale motivo, allora, dobbiamo vincolare burocraticamente l'organizzazione delle unità? I dipartimenti sono l'innovazione principale di questa legge: lasciamoli agire per la creatività della ricerca e della didattica.

mi sembra che il relatore ci abbia spiegato il perché del suo parere contrario sulla questione della proliferazione dei dipartimenti.

Questo non è possibile: visto che il numero minimo è fissato a 35, bisognerà inventarsi sette docenti da trasferire in modo inopportuno in quel dipartimento per raggiungere il numero minimo, con tutta una serie di inutilità e di contenziosi che violano la possibilità di rendere agile, semplificare e sviluppare l'opportunità del merito e nel merito di quei dipartimenti. debbano avere un numero minimo di docenti fa sì che saremo l'unico Paese occidentale in cui gli atenei non potranno avere un dipartimento di lingua e letteratura nazionale. La lingua e la letteratura italiana sono senz'altro una delle eccellenze di cui dispone il nostro Paese e la nostra accademia. Peraltro, ci stiamo avvicinando alla celebrazione celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e la questione dell'Unità d'Italia è strettamente intrecciata alle radici e alla costruzione di un'unità culturale. L'unità culturale italiana è stata sviluppata grazie a quel grande processo, anche istituzionale e politico, che è stata la costruzione di una lingua italiana. Ora, l'unica cosa che forse precede i 150 anni dell'Unità d'Italia è stata proprio la straordinaria avventura della lingua italiana. In altri Stati, la lingua la lingua nazionale è stata l'esito più costrittivo della costruzione del processo dell'unità Stato Nazione. Nel caso dell'Italia, invece, la lingua di Dante precede l'unità nazionale. Noi saremo l'unico Paese dell'Occidente a non avere dipartimenti di italianistica, di lingua e cultura nazionale. Questo è gravissimo, proprio perché è un patrimonio fondamentale, che non solo deve essere soggetto ad una conservazione,

che trattiamo dell'università, ed è anche il sintomo di un difetto di autonomia, che invece dovrebbe essere il principio filosofico cui dovrebbe ispirarsi la riforma dell'università.

«*i-*bis) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca;».

negli esami, delle conoscenze linguistiche. Tutto ciò va in questa direzione. Volevo sottolineare questo aspetto per ringraziare il senatore Rutelli per un'ulteriore spinta in questa direzione, che darà alle università italiane una

è molto più importante accettare quelle modificazioni che non ragionare su questo articolo. Credo che il diritto di un giovane ad esprimere il suo talento debba essere garantito dalla comunità, anche perché è un diritto della comunità non perdere talenti. L'università serve allo sviluppo della persona umana e alla preparazione alla sua futura professione, ma serve anche allo sviluppo del Paese. di sostegno ai meritevoli costituisce anche un diritto costituzionalmente garantito, ma bisogna anche fare in modo che questo diritto, che io chiamo al completamento degli studi - perché certo non è il diritto agli studi in senso stretto abbia una percorribilità che lo renda attuabile. Come era presentato all'inizio nel testo del disegno di legge del Governo, era un articolo evanescente. Noi prevediamo i criteri per individuare la graduatoria nazionale, per garantire l'anticipo semestrale, per portarsi appresso nell'università che si è scelta la propria borsa di studio. Oggi tanti sprechi intellettuali ed economici, anche nell'organizzazione dei corsi e delle lauree, sono legati al fatto che non c'è mobilità nemmeno degli studenti nello scegliersi l'università. Chi è in difficoltà in termini economici, chi non può pagare l'accoglienza abitativa altrove, sceglie l'università più vicina a casa e crea quel circuito vizioso che ha molto danneggiato sia i giovani sia le università. Quindi, questo è un articolo riscritto in modo da rendere vero ciò che forse, nelle intenzioni del Governo, c'era nell'articolo 4. Se il Governo accettasse questo mio emendamento ne sarei onorata, perché vorrebbe dire che in questa

senatore Livi Bacci soprattutto per una legge di riforma dell'università che molto dovrebbe basarsi sulla valutazione. L'ANVUR è una delle sigle più citate. Purtroppo, è anche una sigla per ora fantasma, perché tale Agenzia è al momento un guscio vuoto, non riempito di contenuti.

Occorrono molte risorse per valutare bene: non bastano dei cervelli buoni nel consiglio di amministrazione. Fatta questa premessa, l'emendamento

permetta di valutare il capitale umano, le competenze degli studenti. Questo servirebbe anche per il fondo per il merito ed in parte è contenuto anche nel disegno di legge n. 1905. Questa valutazione all'ingresso, inoltre, deve essere accoppiata ad una valutazione all'uscita dall'università e, quindi, a un test sulle competenze e le conoscenze degli studenti al momento

corso, dalla localizzazione geografica, e via dicendo. Quindi, un test nazionale permette alle varie università di conoscere la qualità del proprio materiale umano. Servirebbe poi all'uscita, perché ci permetterebbe di vedere qual è il guadagno di conoscenza che si realizza nei vari atenei. Faccio un esempio molto semplice. Prendiamo due università, l'università di Castelforte di Sopra e l'università di Castelfranco di Sotto: a Castelforte di Sopra gli studenti, all'entrata, hanno un livello pari a otto e gli studenti all'uscita un livello pari a dieci; quindi, c'è stato un guadagno di efficienza.

premiare di più l'università che ha il livello dieci con i fondi ordinari e che ha guadagnato due, o vorremmo dare più merito all'università di Castelfranco di Sotto

ma a livello di corso di laurea, di università, cioè a livello statistico, il test serve molto a capire la media. Una persona che non è capace a risolvere un cruciverba non è necessariamente un citrullo, può anche essere un genio,

atto della trasformazione in ordine del giorno

Presidente, per rispetto ai tanti cittadini e ai tanti studenti di questo Paese, più che ai professori, penso al miliardo e 300 milioni che mancano a questa università, penso ai 26.000 ricercatori e ai due milioni di studenti, più che all'ordine del giorno. Vorrei quel risultato.

mostrasse più attenzione e un po' più di condivisione verso le richieste che vengono dai cittadini e dalle università italiane, che rappresentano una priorità per questo Paese.

È noto che l'articolo 64 del nostro Regolamento stabilisce, al secondo comma, che il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi con il Presidente della Camera per la convocazione dei senatori.

trascurando anche quel minimo di vettovagliamento che non è negato a nessuno. Detto questo, so che in seconda battuta posso chiedere anche a lei, signor Presidente, se, apprezzate le circostanze, che sono fondanti secondo me, non intenda togliere la seduta.

in un Comune vicino Lucca, dove un dipendente licenziato è entrato nell'azienda presso cui lavorava e ha ucciso due persone, per poi suicidarsi. È un episodio che ha scosso molto l'opinione pubblica italiana. Molto si è parlato delle condizioni personali e dei rapporti di lavoro, come è giusto che fosse. Troppo poco si è parlato di un'altra questione: quell'uomo era un legittimo detentore d'armi. Quella persona era in cura psichiatrica da tre anni nei servizi territoriali del luogo in cui era residente, eppure le autorità preposte al rilascio del porto d'armi non hanno revocato il permesso. Come alcuni colleghi sanno, ho depositato

vittime dovranno ancora esserci, in particolare giovani donne. Questo non è stato che l'ultimo episodio di un mese e mezzo di vittime della follia,

ora, però, che la questione della detenzione di armi da parte di persone con squilibri mentali venga affrontata con grande responsabilità e urgenza: lo dobbiamo alle tante vittime e ai loro familiari!

Ho cercato di informarmi, perché una mostra organizzata in Senato sull'Unità d'Italia, in occasione dei 150 anni dell'Unità stessa, ha indubbiamente una notevole

il quale tra l'altro aggiunge anche i costi per il personale, perché - come è giusto che sia - le sale rimangono aperte anche nelle giornate di sabato e di domenica.

terminando l'esame di una manovra finanziaria notevole, della quale abbiamo dovuto rispondere agli italiani rispetto ad una serie di spese. Credo, dunque, che il Senato debba correttamente rispondere anche di questa spesa.

sostanzialmente uccidendo un'eccellenza della produttività del nostro Paese, cioè l'industria farmaceutica nazionale, e precisamente quella dei principi attivi. L'industria farmaceutica, che esporta

tutte quelle procedure che si adottano per mettere in commercio tonnellate e tonnellate di prodotto. È un'assurdità!